Onorevoli senatori, comunico che nella seduta antimeridiana di domani la sottosegretario di Stato per l'interno, avvocato Viale, renderà un'informativa del Governo sui flussi migratori a Lampedusa. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

basata sull'incenerimento e sulle sue varianti (a cominciare dalla cosiddetta termovalorizzazione) costituisce il problema e non la soluzione di una corretta ed efficace gestione dei rifiuti. La soluzione è invece da rinvenire nella gerarchia di azione stabilita dalle direttive comunitarie di settore, che privilegiano il riciclo, il riuso dei materiali e - a monte - la differenziazione spinta con raccolta porta a porta. Tutto questo, che peraltro è formalmente scritto anche nella legislazione vigente, nella regione che ospita la capitale d'Italia è oggi lontano anni luce dalla sua realizzazione, così come è stato evidenziato dal relatore, senatore De Angelis. Già nel marzo scorso avevamo ben presente il rischio che dal lavoro istruttorio della Commissione bicamerale non potessero emergere adeguatamente le criticità della situazione. Tali dubbi hanno ricevuto una conferma proprio oggi, in quanto la situazione di emergenza ambientale dell'unica discarica operante a Roma da alcuni decenni, quella di Malagrotta, è venuta in evidenza in tutta la sua drammaticità. Occorrerà, in particolare, capire se i dati sull'inquinamento dell'area saranno confermati e, di conseguenza, chiarire come mai essi non siano stati resi noti in passato. La Regione si è dotata, nel novembre 2010, 2010, di un Piano regionale inadeguato, le cui incongruenze più evidenti stanno nella palese irrealizzabilità degli obiettivi prefissati e nella inidoneità dei mezzi scelti per conseguirli, al punto che la medesima Regione ha chiesto la deroga per gli stessi obiettivi. Il ricorso privilegiato allo smaltimento in discarica alla realizzazione di impianti CDR e di inceneritori veri e propri ha determinato - anche nel Lazio - il fallimento della programmazione della raccolta differenziata, perpetuando quel conflitto di interessi che non consente il ritorno ad una gestione ordinaria ed ordinata. dell'Italia dei Valori ritiene - inoltre - che le scelte relative alla localizzazione degli impianti non possano più essere calate dall'alto sulle comunità locali e sulle autonomie territoriali - soprattutto - imposte senza tenere in considerazione tutte le possibili alternative, per di più con procedure derogatorie in materia di VIA, di tutela della salute pubblica e di salvaguardia delle risorse idriche. Il recente Piano regionale di gestione dei rifiuti rischia quindi di riproporre nel Lazio il quadro desolante che si registra nelle maggiori regioni del Sud, con il corollario di costi elevatissimi, servizi inefficienti e discariche al collasso, ma prorogate in deroga alla normativa vigente. In molti comuni della provincia di Roma (con l'eccezione della capitale) la raccolta differenziata funziona. Se, però, si continuerà a puntare sull'impiantistica tradizionale e ad ignorare il compostaggio, ogni sforzo sarà vano, poiché Roma produce da sola quasi i due terzi dei rifiuti regionali. La risoluzione proposta all'Assemblea ha rilevato le criticità che ho appena indicato ed ha anche evidenziato il rischio serio ed incombente di penetrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti della Regione. Non è solo la vicinanza geografica con alcune zone della Campania a determinare tale rischio. Il Lazio è la seconda regione d'Italia per PIL prodotto dopo la Lombardia ed una delle prime per prodotto interno lordo *pro capite*; è una regione che vede proprio nella zona di Roma la massima produzione di reddito nel settore dei servizi. È dunque illogico ipotizzare che le varie mafie non abbiano come obiettivo la penetrazione territoriale in questa regione e dalla Commissione antimafia sappiamo - infatti - in quali aree già si sono installate organizzazioni criminali di origine calabrese, siciliana e campana. In questo quadro, l'impiantistica pesante è da sempre l'obiettivo dei finanziamenti e delle agevolazioni amministrativo-burocratiche e - dunque - esercita un'attrattiva per la criminalità ambientale ed economica. Al contrario, la carenza di fondi affligge l'apparato istituzionale di controllo (magistratura e forze dell'ordine in primo luogo), chiudendo in tal modo un circolo vizioso, in cui rischi di infiltrazione mafiosa, inefficienza della macchina pubblica, situazioni di monopolio di fatto e distorsioni del mercato, regime derogatorio e minor trasparenza delle procedure producono invariabilmente un aumento dei costi a carico dei cittadini. L'impegno che chiediamo al Governo è anzitutto quello di reperire idonee risorse per il presidio del territorio e per le forze dell'ordine in particolare, e di non indebolire gli strumenti investigativi e i mezzi di indagine. L'impatto che i disegni di legge sulle intercettazioni, sulla prescrizione breve e sul processo lungo avrebbero sui reati ambientali - compresi, quindi, anche quelli relativi alla gestione dei rifiuti - è evidente.

recuperare le materie: le cosiddette «quattro erre») devono costituire il primo ed essenziale campo di collaborazione tra istituzioni nazionali e regionali. In tal senso, ci rallegriamo del fatto che il Governo abbia fatto marcia indietro sull'abrogazione del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) e che il Ministro dell'interno abbia duramente censurato l'ipotesi del suo collega Brunetta sulla certificazione antimafia, inducendolo ad una rettifica. Ma questi sono solo i maggiori danni evitati. Quel che manca è la buona amministrazione ordinaria. Né il sindaco della capitale, né la Regione hanno un piano credibile. Non esistono, rispetto allo smaltimento di Roma, alternative serie. Non c'erano a marzo e tuttora non si è riusciti a crearne. A dispetto di ogni campagna pubblicitaria, nella capitale del Paese ancora domina la raccolta indifferenziata: il rifiuto viene sotterrato e il percolato si diffonde.

Le esperienze positive in Italia e all'estero non mancano: è quindi opportuno che il Lazio e Roma in particolare prendano esempio da queste eccellenze e ad esse si adeguino. Con tale imprescindibile premessa, il voto dell'Italia dei Valori sulla risoluzione che censura la gestione dei rifiuti nella Regione Lazio è favorevole.

il diritto alla salute, la lotta alla criminalità organizzata, la salvaguardia del decoro urbano. Tale intreccio, oltre a rendere particolarmente complessa e delicata la gestione della materia, favorisce la cattiva abitudine italiana di demandare altrove le proprie responsabilità, ossia genera un vergognoso scaricabarile. Come ha ben documentato la relazione che oggi discutiamo, il problema rifiuti nel Lazio non è meno grave di quello campano e siciliano, laddove la formale cessazione della gestione emergenziale nell'anno 2008 non ha corrisposto affatto al superamento delle gravi criticità in corso. Il Lazio, con il 9 per cento della popolazione nazionale, produce il 10 per cento dei rifiuti italiani e non ha ancora attivato tutte quelle procedure di ammodernamento cui ricorrono, anche a fronte di numeri meno importanti, i Paesi più avanzati d'Europa. A ricordarcelo vi è l'attivazione di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea, che domani, come è noto, deciderà se mettere in mora l'Italia per l'emergenza rifiuti di Napoli. Lo scempio della capitale partenopea, cui più volte abbiamo assistito negli ultimi anni, si ripeterà anche a Roma e in altre città del Lazio se non si correrà immediatamente ai ripari. Tra appena due mesi, il 31 dicembre - lo ha detto il chiuderanno i cancelli di Malagrotta, la storica discarica che per trent'anni ha inghiottito tutti i rifiuti della capitale, e sarà piena emergenza. Ma cosa si sta facendo per evitare questo disastro annunciato? Nulla di concreto. Un dato per tutti: la raccolta differenziata nel 2010 si è attestata su valori del 12-13 per cento. Il nuovo piano di gestione dei rifiuti del novembre 2010

Da qualsiasi prospettiva si guardi al problema, la percezione è sempre la stessa: il tempo è scaduto. Occorrono, infatti, almeno tre anni per la realizzazione di una nuova impiantistica prevista dal Piano e quattro per l'attivazione di una nuova linea di termovalorizzazione. Così, nel frattempo, si ricorre all'unica strada abbandonata da tutta Europa, quella delle discariche; e con molte difficoltà, perché non sappiamo ancora dove verrà aperto il nuovo invaso, dato che si sta delegando il problema ai privati, col rischio di mostruose speculazioni. Tutto ciò naturalmente è terreno più che fertile per le ecomafie. Anche oggi ho sottolineato questo aspetto in Commissione antimafia al Prefetto ed al Questore, invitati per una audizione, evidenziando la possibilità che la mafia metta le mani su questo problema. La relazione oggi alla nostra attenzione ha rilevato con allarme gli illeciti accertati nella gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Colleferro, illeciti favoriti dalla carenza nel sistema di controlli da parte di Comune, Provincia e Regione. Il Lazio, come segnala ancora la relazione, si presta fin troppo bene alle infiltrazioni della criminalità in questo settore, sia perché territorio adatto alla discarica e all'occultamento dei rifiuti, sia per la sua prossimità con quelle aree della provincia di Caserta dove le ecomafie prosperano da tempo. E non è una novità: in località quali Cassino, Pomezia, Latina, Formia e Ardea sono 40 anni che si riscontrano insediamenti della criminalità organizzata siciliana, calabrese, ma soprattutto campana. Sul piano sanitario, un dato per tutti è esemplificativo delle proporzioni dell'emergenza: è in corso un'inchiesta per omicidio colposo su quattro morti di tumore tra gli abitanti dei dintorni di Malagrotta.

È tempo dunque di passare dalle parole ai fatti; è tempo che qualcuno si faccia carico sul serio di questa situazione. Sulla base della relazione in esame, largamente condivisa in Commissione, la parte politica che rappresento chiede con forza che quest'assunzione di responsabilità venga prima di tutto da parte del Governo sotto forma di un piano serio e tempestivo per attuare le bonifiche. Realizzare bonifiche vuol dire dare fiducia ai cittadini, vuol dire recuperare credibilità da parte della politica e vuol dire dimostrare che si ha cura della salute dei cittadini e la si ha a cuore. Solo riconquistando la fiducia infatti, potremo poi chiedere loro di appoggiare le grandi scelte in tema di localizzazione e la realizzazione degli impianti di trattamento. Auspichiamo dunque, signora Presidente, che questo Parlamento dilaniato dalle divisioni possa oggi, su un tema così delicato e in presenza di una relazione approvata all'unanimità, dare finalmente l'*input* necessario a mettere mano a una situazione che degenera di ora in ora.

onorevoli senatori, dalla relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e dal dibattito svolto in Aula è emersa chiaramente una drammatica analogia di scenari e di criticità tra ampie aree del Sud del Paese in tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. La regione Campania fa da capofila, ma seguono le realtà della Sicilia e del Lazio. L'eccellente lavoro d'indagine svolto dalla Commissione d'inchiesta ha messo in rilievo una situazione disastrosa per la regione Lazio. L'emergenza rifiuti perdura sin dal 1999; la gestione commissariale, formalmente, è cessata nel 2008, ma le criticità ancora permangono; l'85 per cento dei rifiuti urbani va ancora in discarica, quella di Malagrotta,

mentre doveva raggiungere almeno il 60 per cento nel 2011. A tutto ciò si aggiungono le debolezze del sistema di controllo e le connessioni tra attività imprenditoriali e fenomeni di corruzione della pubblica amministrazione. Dall'analisi svolta dalla Commissione sembra che i cittadini di Roma corrano il serio pericolo di trovarsi a breve in una condizione identica Lo scenario è preoccupante e perciò occorrono interventi immediati da parte delle amministrazioni, evitando lo scarico di responsabilità tra amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra, tra Comune e Regione. Non voglio ripetere per l'ennesima volta gli esempi virtuosi del Nord, ove i Comuni già da decenni attuano la raccolta differenziata, arrivando a risultati superiori all'80 per cento di materiale differenziato. La spaccatura del Paese nella gestione dei rifiuti è oramai nota a tutti: la raccolta differenziata supera la media nazionale e per la parte indifferenziata ci sono i termovalorizzatori; al Centro-Sud mancano sia la differenziata che i termovalorizzatori. Penso tuttavia che tutti convengano come la situazione del Lazio sia dovuta ad una cattiva amministrazione, ad una mancata previsione e a carenze che hanno origini in anni addietro e non dipendono solo dall'amministrazione attuale. Il nostro Gruppo nella Commissione bicamerale ha votato il documento conclusivo, anche perché occorre far emergere il lavoro responsabile svolto dalla Commissione, occorre elogiare i 12 anni di attività ispettiva svolta dalle forze dell'ordine, in particolare dai Carabinieri e dalla Guardia di finanza. La Lega Nord ha sottoscritto la risoluzione e voterà a favore (come già avvenuto alla Camera), sollecitando tuttavia le amministrazioni locali e regionali ad individuare soluzioni immediate per fare fronte alle criticità e per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche emerse, puntando soprattutto, con un rinnovato spirito federalista, all'aumento di responsabilità da parte degli amministratori. Da parte sua la Commissione bicamerale dovrà continuare il lavoro di controllo e di monitoraggio, connesso sia agli sviluppi legati alle infiltrazioni della criminalità organizzata, sia ai fenomeni di corruzione della pubblica amministrazione che sono stati evidenziati nelle indagini svolte. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

rispetto agli illeciti nel ciclo integrato dei rifiuti, per rassegnare all'Aula del Senato una valutazione rispetto alla opportunità che questa Commissione offre al Parlamento,

che questa Commissione ha verificato attraverso audizioni e sopralluoghi sul territorio nazionale, dove purtroppo non c'è solo un ritardo della della politica riguardo al tema del ciclo integrato dei rifiuti rispetto alle direttive europee, ma c'è una presenza drammatica

che non ha subito nessuna crisi, nessun rallentamento ed è quello dell'ambiente, quello della salvaguardia del territorio, che è anzi una possibilità di crescita

Stiamo lavorando in questo settore su una legge quadro rispetto al ciclo integrato dei rifiuti. La vicenda dalla regione Lazio accumula - ahimè! - drammatici ritardi. Non si può vivere solo di discariche e di commissari *ad acta*,

tentare di evitare i rischi pericolosi dal punto di vista non solo di una aggressione delle mafie - per dirla con Pietro Grasso, procuratore distrettuale antimafia

i rifiuti sono una straordinaria risorsa che non può essere dispersa. Credo che questa possa essere una occasione, anche rispetto all'ultima manovra del Governo,

di oltre 200 cave abbandonate, piene di rifiuti industriali che devono essere bonificate (ed è questo un altro settore totalmente dimenticato).

impone anche, in qualche modo, un indirizzo dal punto di vista della direttiva europea. Non è possibile un contrasto tra lo Stato e le Regioni e spesso - come è capitato nell'emergenza

Come si può immaginare, anche solo per un attimo, di eliminare la tracciabilità dei rifiuti abrogando il SISTRI, quando l'Europa ce lo chiede? Come si può immaginare - come ha detto qualche Ministro - di eliminare i certificati antimafia? In questo modo facciamo un regalo senza freni alla malavita organizzata,

da parte del Parlamento, delle forze politiche e da parte dei cittadini. Il ciclo integrato dei rifiuti crea una condizione virtuosa, di crescita di civiltà e anche di sviluppo, che non possiamo abbandonare.

fatto comprendere il lavoro attento che la Commissione ha svolto in questo campo: un lavoro che si è protratto con gli incontri e le audizioni con le autorità responsabili. Ha fatto bene il collega relatore a ricordare che il prefetto di Roma è responsabile, per delega del Governo, del problema della discarica

ha avuto e ha, proprio in questo territorio, responsabilità politiche e amministrative. Sarebbe facile per me tornare un attimo indietro, senatore De Angelis, sulle responsabilità di un piano mai attuato, di impegni mai presi, di responsabilità scaricate tra Regione e Comune, tra opposizione e comitati, perché ogni volta che si parla di questo problema, siamo tutti d'accordo che nessuno vuole la discarica nel proprio giardino, ma nessuno vuole che i rifiuti

che ha avuto in questi anni, ha retto alle necessità di una grande città come Roma e anche dei Comuni limitrofi. Sappiamo perfettamente che è difficile trovare i modi e i termini per convincere gli amministratori locali ad avere nel proprio territorio delle discariche o degli impianti. Il problema è sempre lo stesso, e al riguardo dobbiamo sottolineare gli aspetti che la relazione della Commissione ha evidenziato, i pericoli che ci sono in questo campo. In quest'ambito, anche negli anni passati ci sono state delle responsabilità, delle inchieste, che hanno dimostrato come le infiltrazioni che vengono dal Meridione siano arrivate nel Sud del Lazio e poi si siano ampliate proprio nel territorio laziale. Ci sono state denunce e una serie di precisi

sicuramente fermato il tentativo di infiltrazione. Tutti sanno che questi tipi di infiltrazione hanno vogliono avere un rapporto con la politica, con la politica del territorio, per andare incontro alle proprie esigenze; esigenze che poi sono fuori dal desiderio dei cittadini di vedere risolto il problema.

un lavoro attento e responsabile da parte degli amministratori dei grandi centri (penso alla città di Roma, alla grande azienda AMA):

questa Commissione l'ha fatto con capacità e all'unanimità) qualsiasi forma di infiltrazione di carattere mafioso, per raggiungere anche un risultato concreto. Il Lazio ha bisogno di questo piano e ha bisogno di risposte precise, e queste risposte non possono nascere da una contrapposizione tra Comuni ed enti locali, tra enti locali e Regione.

Onorevoli colleghi, informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 28 settembre, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la circoscrizione Estero-ripartizione America meridionale: Esteban Juan Caselli e Mirella Giai. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, all'articolo 6, comma ha delegato il Ministero della difesa a rideterminare con proprio decreto il canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa. L'amministrazione della Difesa ha un patrimonio immobiliare ad uso abitativo di circa 18.500 alloggi dislocati sull'intero territorio nazionale. Circa 5.000 alloggi sono utilizzati da utenti cosiddetti *sine titulo*, ovvero da personale in quiescenza che corrisponde un canone fissato annualmente dal Ministero della difesa, che da tali canoni raccoglie circa 35 milioni di euro l'anno. Va specificato che gli utenti senza titolo concessorio godevano della normativa prevista dalla legge n. 537 del 1993 (articolo 9, comma 7) e dalla legge n. 724 del 1994 (articolo 43). Queste leggi prevedevano che, con decreto annuale del Ministero della difesa, fossero stabiliti i redditi entro i quali si poteva usufruire dell'equo canone e quelli per cui c'era una maggiorazione del 50 Non si tratta dunque di occupanti abusivi, ma di utenti con regolare contratto registrato, che pagano regolarmente l'affitto, e a cui l'importo dovuto per il canone di affitto, stabilito annualmente con decreto ministeriale, viene direttamente detratto dallo stipendio, quindi direttamente alla fonte. Parliamo di militari o comunque di personale in forza al Ministero della difesa, che ha servito lo Stato durante la sua vita. Il Ministero ha recepito la delega e il 27 maggio ha emanato il proprio decreto. Ad oggi, però, il Ministero non ha ancora determinato i nuovi canoni di mercato, considerata anche la difficoltà oggettiva dovuta all'elevato numero di alloggi e la difficoltà di ottenere le quotazioni immobiliari OMI. Per questo il Ministero ha avviato una procedura che vorrebbe applicare un canone di mercato provvisorio, salvo poi conguaglio all'atto dei conteggi parametrali veri e propri. È di tutta evidenza che si tratta di un artifìcio, per non dire abuso, che nulla ha a che vedere con quanto previsto dal regolamento dei canoni di mercato. Va detto che parte degli alloggi a cui si chiede che vengano applicati i canoni di mercato sono in condizioni di elevato degrado, per non dire fatiscenti. Personalmente ho avuto occasione di vedere alcune di queste case e non sono rari i casi in cui sono evidenti infiltrazioni, crepe sulle pareti, muri privi di intonaco; in alcuni casi sono visibili ponteggi che da anni sorreggono muri o tettoie pericolanti,

Dall'ultimo decreto del Ministero della difesa sono stati individuati 3.022 alloggi da alienare. La vendita però non sarà approvata prima di due anni. Intanto, gli affitti aumentano. Va, inoltre, ricordato che l'ultima legge finanziaria ha previsto che, in caso di dismissione degli immobili, il ricavato della vendita sarà assegnato solo in minima parte al Ministero della difesa. Come è ovvio, se queste risorse arrivassero per intero al comparto della Difesa, sarebbe possibile investirle, soddisfacendo, così, sia le richieste dei giovani militari che sono in attesa di un alloggio sia quelle dei *sine titulo*. Inoltre sarebbe opportuno attuare il programma pluriennale per la realizzazione, la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate, da tempo predisposto. Va poi detto Va poi detto che parte del patrimonio della Difesa non è stato messo in vendita perché alcuni immobili non sono stati accatastati; in alcuni casi essi risultano sconosciuti al catasto, in altri sono accatastati per uso non abitativo. Basti pensare che metà degli alloggi presenti alla Cecchignola, all'interno della città militare di Roma, non è accatastata. A riprova di ciò, nessun alloggio della Cecchignola è in vendita. Per questo, con la mozione, chiediamo al Governo che vengano individuati a breve termine altri alloggi da alienare, anche risolvendo i contenziosi in essere. Inoltre chiediamo che venga fatta una miniproroga e venga sospesa ogni eventuale azione finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio. La legge n. 244 del 2007 assicura la permanenza per gli affittuari con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale e tenendo conto della presenza di portatori di handicap tra componenti del nucleo familiare. Il regolamento attuativo invece circoscrive a cinque o sette anni la permanenza e riduce sensibilmente il reddito familiare lordo complessivo, portandolo a soli 19.000 euro annui. Inoltre, l'usufrutto non è più il rischio è quello di mandare via i vecchi inquilini, che hanno regolarmente pagato il canone di locazione, per trovarsi con appartamenti vuoti. Inoltre, nella nuova normativa che disciplina i canoni e le vendite, viene introdotto un metodo piuttosto bizzarro. Per calcolare il canone di locazione, infatti, oltre al reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, è aggiunto un fantomatico coefficiente correttivo calcolato in base al periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo concessorio. Che è un po' come dire: «avevate per legge tutti i diritti per abitare in quelle case, avete pagato regolarmente l'affitto, ma ora ci dovete ridare indietro un po' di soldi». Nei contratti di locazione privati, gli aggiornamenti , avvengono automaticamente al 75 per cento. Ciò accade anche per i senza titolo concessorio, ma gli adeguamenti sono al 100 per cento degli aggiornamenti ISTAT. Tutto ciò può essere sufficiente per spiegare una situazione che è di fatto difficilissima e che rappresenta un accanimento senza senso da parte del Ministero della difesa. Con la mozione, quindi, chiediamo di sopprimere le norme contenute nel regolamento vendite, articolo 7, punto 11 e le norme previste all'articolo 2, del decreto ministeriale 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato, e di ricondurre al 75 per cento la norma relativa all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione annuale. Inoltre, chiediamo, vista la condizione di alcune abitazioni, in caso di assegnazione di alloggio o in caso di lavori di manutenzione di un alloggio occupato, la possibilità, con il tassativo consenso delle parti, di far eseguire i lavori a spese dell'inquilino, prevedendo la detrazione delle spese sostenute dal canone di affitto. In conclusione, con la nostra mozione non chiediamo di salvaguardare una determinata categoria di cittadini, bensì chiediamo all'amministrazione quella coerenza amministrativa, procedurale e normativa, unita alla salvaguardia delle esigenze di economicità, efficacia e trasparenza pubblica, che dovrebbero essere alla base del nostro dettato costituzionale

la mozione n. 467, a prima firma del senatore Scanu, sugli alloggi di servizio per i militari, attiene ad una problematica di grande delicatezza e complessità: concerne infatti le aspettative coltivate da tutto il personale militare nei confronti di un bene essenziale: la disponibilità di un alloggio per la propria famiglia durante il servizio attivo e dopo la sua conclusione. Ho parlato di tutto il personale in uniforme: le misure promosse nel settore degli alloggi militari non possono infatti, a mio avviso, essere destinate a soddisfare le esigenze solo di una parte di quel personale, ma devono rivolgersi a tutta la categoria. Devono essere indirizzate decisamente e efficacemente verso i militari in servizio, quelli che garantiscono con la loro attività e la loro professionalità l'assolvimento dei compiti della difesa e della sicurezza nazionale. Ma devono rivolgersi anche al personale meno giovane e non più in servizio attivo, personale che, non dobbiamo dimenticarlo, ha operato per decenni con le stellette per il bene della Patria e la crescita delle istituzioni. Tutti, gli uni e gli altri, hanno svolto in passato o stanno svolgendo attualmente una funzione caratterizzata da dedizione, sacrifici e continua disponibilità, una funzione che finalmente in questa legislatura ha avuto un riconoscimento formale con la definizione della loro specificità di impiego. Non è facile trovare immediatamente soluzione alla problematica degli alloggi per i militari: basti considerare la grande differenza esistente tra la disponibilità, che attualmente ammonta a circa 18.000 alloggi, e le molte più numerose esigenze degli appartenenti alle Forze armate, ormai tutte La mozione n. 467 evidenzia quindi degli aspetti che consentirebbero, se posti in essere, di modificare in senso positivo la situazione in questo settore. La prima sollecitazione che la mozione rivolge al Governo è finalizzata a sostenere le aspettative del personale in servizio, che chiede giustamente di svolgere i propri delicati compiti senza essere condizionato da problemi di sistemazione alloggiativa per sé e la famiglia.

quel programma che è stato avviato con la finanziaria 2008, approvata nella precedente legislatura, nella consapevolezza che le esigenze alloggiative degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari destinati destinati a permanere nelle strutture della Difesa per l'intera vita operativa possano essere soddisfatte solo grazie ad un progetto di grande impatto e di consistente durata, capace conseguentemente di risolvere il problema della casa in forma completa. La mozione impegna il Governo anche a incrementare sensibilmente il numero delle strutture non più essenziali per le esigenze della Difesa, che possono essere messe in vendita per realizzare con le risorse ricavate nuovi e più funzionali alloggi; quelli finora individuati per l'immissione sul mercato, poco più di 3.000, costituiscono solo il primo insufficiente blocco. La mozione del Partito Democratico, in armonia con i suoi obiettivi, rivolge una forte attenzione anche all'altra parte del personale militare, quello non più in servizio, che occupa ancora alloggi militari e che non può essere trascurato trascurato dalla politica perseguita dall'Esecutivo in questo settore. Innanzitutto, per il periodo di rivitalizzazione del programma pluriennale che ho prima ricordato e che darebbe soluzione alla problematica della disponibilità di alloggi, evidenzia l'opportunità della sospensione dei recuperi forzosi delle abitazioni eventualmente già disposti. Rivolge poi la sua attenzione proprio verso i rapporti con i conduttori di alloggi militari che hanno lasciato il servizio attivo senza prevedere per essi alcun particolare privilegio, ma solo l'attuazione nei loro riguardi delle tutele già previste da norme di legge per gli utenti titolari di un reddito compreso in fasce protette. Tra le citate tutele, sottolineo il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per gli inquilini che non siano in grado di acquistarlo, qualora l'alloggio stesso sia posto in vendita nell'ambito del programma pluriennale; pluriennale; il diritto alla permanenza negli alloggi dei conduttori e del coniuge superstite con basso reddito o con componenti portatori di *handicap*; di *handicap*; il diritto del conduttore di vedersi attribuito un canone di affitto dell'alloggio congruo con il suo reddito reale; il diritto, infine, di vedersi applicato nel canone l'aggiornamento annuale l'aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 75 per cento, entità normalmente applicata per i canoni privati, anziché nella ingiustificata misura del 100 Sono semplici esigenze di carattere sociale quelle evidenziate dalla mozione ed il loro mancato accoglimento sarebbe sicuramente interpretato come scarsa attenzione nei confronti del personale in quiescenza e delle sue famiglie. In sostanza, la mozione affronta una tematica che merita un esame approfondito e condotto con equilibrio. Mal si prestano, a mio avviso, su questo argomento le assolute certezze e le decisioni non attentamente ponderate. Sia le une che le altre rischiano di non focalizzare al meglio gli aspetti sociali della problematica e le difficoltà che possono derivare, nelle persone e nei nuclei familiari, dalla fredda applicazione di norme rigide e talvolta percepite come inique. C'è bisogno quindi di un confronto aperto che non può essere limitato ai lavori odierni di quest'Aula. Un confronto che deve allargarsi ed approfondirsi, considerato anche che, solo nella giornata di ieri (e quindi dopo la presentazione delle mozioni), la problematica degli alloggi per il personale non più in servizio è stata riproposta nel contesto di un nuovo schema di decreto legislativo all'attenzione ora della Commissione difesa e concernente modifiche al codice dell'ordinamento militare. In questo quadro ed in considerazione dell'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla delicata tematica in esame, chiedo che, una volta conclusa la fase di illustrazione delle mozioni presentate, ne sia rinviata la discussione. Ciò al fine di consentire alla Commissione di merito, attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento ed i contributi dei rappresentanti del personale interessato alla questione, un supplemento di esame esame per giungere, auspicabilmente, ad un testo pienamente condiviso da tutte le parti politiche.

vorranno ascoltarmi e sono interessati sulla realtà che contraddistingue questo problema. Come è stato accennato, la disponibilità di alloggi dell'amministrazione della Difesa per i suoi appartenenti

disponibili e più di 50.000 richieste). A quel tempo, così come oggi, il Ministero della difesa, preso atto di questa carenza, definì i criteri per l'assegnazione degli alloggi e i tempi in cui potevano essere occupati. Non avendo tanti alloggi quanti i richiedenti, ovviamente si pensò di ridurre i tempi di fruizione e si definirono in quattro o otto anni, dopo di che si doveva lasciare posto ad altri che avevano analogo diritto. Ad un certo punto, alcuni cominciarono a non uscire più dopo quattro o otto anni e allora il Ministero, come stabilito per legge, iniziò le procedure di sfratto. Fu in quel momento che scoppiò il pasticcio, perché, da parte del Parlamento, alcuni zelanti, citando certe ragioni che ho sentito riecheggiare anche oggi, sospesero l'azione di sfratto

5.000 senza titolo, che hanno danneggiato 15.000, 20.000 o 30.000 che, con analogo diritto, non hanno potuto usufruire di questi alloggi. Questa è la verità. è la verità. Come è stato ricordato, la situazione è molto ingarbugliata proprio a causa degli interventi irresponsabili dei parlamentari, i quali sono riusciti, in più riprese, a sospendere sempre l'azione di sfratto. Nei confronti di chi? Nei confronti di chi abusivamente è rimasto dentro. Costoro affermano anche di pagare l'affitto e, quindi, di avere un diritto. Ci mancherebbe pure che fossero abusivi e non pagassero neanche l'affitto! manovra finanziaria per il 2008 è stata indicata la necessità e delegato il Governo ad avviare un programma di ricostruzione di nuovi alloggi (anche tenendo conto della variazione dello schieramento delle forze in Italia, il variare della minaccia e della necessità di sicurezza) attraverso la vendita degli alloggi non ritenuti più necessari, la vendita degli alloggi occupati abusivamente (a meno che gli occupanti non vogliano acquistarli, favoriti anche da diminuzioni di prezzo) e, poi, la costruzione di nuovi alloggi. Il Ministero ha svolto le procedure - non facili - e oggi è già in condizione di iniziare la vendita. del Popolo della Libertà presenta una mozione che prende atto di tutti i passi che sono stati fatti, quali il Programma e la definizione del regolamento e degli alloggi che possono essere venduti. però, dal momento che il discorso parte dal 2008 e siamo già nel 2011, la mozione sollecita, incita e stimola il Governo a dare attuazione a quanto previsto, preso atto che sono state svolte tutte le procedure e tutti i passi per cominciare a realizzare il programma. Il Gruppo del Popolo della Libertà chiede pertanto al Governo di portare rapidamente a conclusione le procedure di alienazione degli alloggi non più utili già individuati,

dagli articoli 401 e 402 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'attuazione del richiamato Programma nei tempi previsti dallo stesso;

ancora una volta (anche se se ne è sempre tenuto conto), delle prioritarie esigenze istituzionali e, contemporaneamente, delle situazioni oggettive, in termini reddituali e familiari, dell'utenza di fatto interessata da tale procedura. Voglio ricordare che sia nella normativa della manovra finanziaria del 2008, sia nei successivi passi svolti dal Governo, si è sempre tutelato il personale protetto: vedove, famiglie con handicappati e altre situazioni che effettivamente meritano considerazione. Ma voglio anche ricordare che molti di questi alloggi sono occupati da persone che non vivono affatto in condizioni precarie. Voglio anche ricordare che il permanere di queste persone in quegli alloggi va a danno - lo dico a chi ha sottolineato la necessità di tenere conto di tutto il personale di tante persone che avrebbero lo stesso diritto, ma che per 10, 20, 30 anni sono rimasti fuori perché questi alloggi sono occupati abusivamente.

di ridiscutere l'argomento, approfondendolo e sperando di riuscire anche a giungere ad una soluzione concordata. A noi questa proposta va benissimo, luogo perché in questo modo non si creano intralci al Governo, che può continuare a procedere nel senso che noi indichiamo; in secondo luogo perché una soluzione condivisa in ambito parlamentare è sempre da auspicare

Signor Presidente, colleghi, illustro molto sinteticamente il documento presentato, a mia prima firma, dal Gruppo Italia dei Valori. Vorrei precisare che si tratta di porre fine ad un problema che è purtroppo fortemente rappresentativo ed emblematico - oserei dire - del modo di gestire la cosa pubblica nel nostro Paese. Il problema di cui parliamo, nella sua complessità, è molto, molto semplice. Ci sono tanti alloggi di proprietà della Difesa: alloggi non tutti caratterizzati, per la Difesa, da una certa utilità; alloggi per la quasi totalità occupati; alloggi, per una percentuale spaventosa (circa un terzo), occupati dai cosiddetti *sine titulo* (tra questi, oltre la metà, non ricadenti nelle fasce cosiddette tutelate). Mi rendo conto che in ballo ci sono stati e ci sono interessi finanziari importanti, ma non si può pensare di mantenere in piedi una situazione del genere. Spero che almeno oggi non si decida per il mantenimento di tali interessi e che si prendano degli impegni precisi. Impegni che per l'Italia dei Valori significano: eliminazione delle iniquità introdotte in tema di concessioni di usufrutto, canoni di mercato, attraverso l'abrogazione dei parametri di cui all'articolo 2, del comma 3, lettera *b),* del decreto ministeriale del 16 marzo 2011; abrogazione di tutte le parti dell'articolo 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 112 del 2010, di fatto in contrasto con le vigenti norme in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione; fare in modo che le variazioni di canone abbiano efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato, e non efficacia retroattiva;

Inoltre, ci auguriamo si voglia adottare ogni altra possibile iniziativa di sostegno agli utenti degli alloggi del Ministero della difesa e recepire le richieste di tutte le associazioni rappresentative degli utilizzatori degli stessi immobili,

discussione per affrontare questa tematica che, come abbiamo potuto vedere, è molto complessa e necessita di approfondimenti e di un confronto ulteriore.

oggi non c'erano le condizioni per la presenza in Aula del Ministro e che avremmo tutti l'intenzione di arrivare a una mozione condivisa,

colleghi, poiché la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non ha concluso l'esame dei documenti all'ordine del giorno, la relativa discussione in Assemblea, prevista per la seduta antimeridiana di domani, non avrà luogo.

c'è una vostra collega che sta intervenendo.

Nata a Milano nel 1921, fu una militante antifascista, iscritta da giovane al Partito Comunista; partigiana, guidò i moti insurrezionali dell'aprile

lei, insieme a Gina Bianchi, detta Lia, che morì il 24 aprile, mentre aspettava un bimbo e mentre correva insieme appunto a Lalla (questo era il nome di battaglia

tra le lavoratrici e in difesa di tutte le battaglie di emancipazione delle donne. Fu la prima donna ad entrare nella segreteria della Camera del lavoro di Milano,

che è tramontata insieme al secolo scorso, ma ha condotto tutta la sua vita all'insegna di una grandissima umanità e soprattutto in difesa, sempre e comunque, delle donne: dalle braccianti del cremonese